Signor Presidente, vorrei rivolgerle un'istanza sull'ordine dei lavori. Come sappiamo tutti, le Commissioni riunite 1ª, 5ª e 6ª stanno esaminando l'importantissimo provvedimento sul federalismo fiscale si trovano nella fase conclusiva dei lavori: oggi devono essere esaminati e votati gli emendamenti al testo che il Comitato ristretto ha predisposto. Poiché è stata convocata una seduta pomeridiana delle Commissioni riunite stesse alle ore 14 e considerando che il nostro Gruppo ha la necessità di assumere un orientamento conclusivo sull'atteggiamento da tenere sul provvedimento, anche alla luce dell'evoluzione di queste ore sulla definizione del testo e degli emendamenti, attività che sono in corso, le chiedo a nome del nostro Gruppo

Nelle more, mentre deliberavamo questo, è arrivato un appunto delle tre Commissioni che all'unanimità chiedevano alla Conferenza dei Capigruppo di non tenere Aula nel pomeriggio di oggi. Ne abbiamo preso atto, visto che la richiesta era formulata all'unanimità dalle tre Commissioni, abbiamo preferito, cambiando percorso di scelte, di non tenere seduta nemmeno nel pomeriggio di oggi e di prevedere la seduta antimeridiana Prendo atto dell'esigenza che mi manifesta a nome del suo Gruppo: la Presidenza è sempre sensibile alle richieste che vengono formulate dai Gruppi per esigenze di riunioni interne. La pregherei di accettare la controproposta della Presidenza di concludere la seduta alle ore 13, anziché alle 13,30, e consentire all'Aula di lavorare su questo importante disegno di legge che - come lei noterà - non è contingentato nei tempi. Vi è un dibattito ampio, serrato e costruttivo Grazie

apre una nuova finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Colleghi, vi pregherei di prestare maggiore attenzione agli interventi dei senatori. Il senatore Li Gotti sta ponendo un problema sull'ordine dei lavori attinente all'argomento in trattazione in

ha dimostrato di saper bene interpretare ed applicare l'articolo 8 del Regolamento relativo all'esercizio dei suoi poteri, mi appello proprio a questa sua

Il costo indicato si rinviene nella relazione tecnica allegata al disegno di legge e viene rapportato

questo cambia notevolmente i numeri della platea dei destinatari dell'intervento. Il Servizio del bilancio del Senato aveva sollevato questo problema, ponendo l'enorme differenza tra i due numeri (49.000 in un caso, 700.000 nell'altro), però ha valutato sulla base dei 49.000, perché quella era quella era la platea interessata dall'articolo 9. Ora però la platea è cambiata, quindi torniamo a quei numeri diversi. L'emendamento L'emendamento presentato dal Governo ha modificato la norma sulla copertura finanziaria, non nelle cifre, che sono rimaste identiche

Sulla base di questa difettosa comunicazione, perché non bastava cambiare il numero dell'articolo,

piccole modifiche, di recepimento delle indicazioni di copertura finanziaria: 33.354.000 euro previsti nel disegno di legge; 33.731.000 euro proposti dalla Commissione bilancio. È la medesima somma, in sostanza. Il problema che io pongo non è di lieve entità. Calcolare il costo dei processi per 49.000 persone porta ad un risultato; calcolare il costo dei processi per 500.000 persone, quanto è la platea dei destinatari di questa norma, significa moltiplicare per dieci la copertura prevista. Significa cioè passare da una copertura di 33 milioni di euro, solo per i processi, ad una copertura che sfiora i 400 milioni di euro. di euro. Se noi manteniamo e prevediamo la copertura così come era originariamente prevista creiamo un grosso problema, perché poi dovremo pagare gli interpreti e gli avvocati per il gratuito patrocinio. Tutti quei costi, stimati per singolo processo in 650 euro dal Ministero, dovremo dunque moltiplicarli e trovare

la concreta copertura finanziaria di questa legge. La ringrazio estremamente articolate, importanti ed interessanti, che hanno una base logica e anche finanziaria.

con un emendamento aggiuntivo al testo iniziale, dei soggetti destinatari di sanzioni penali e quindi di procedimenti penali, per cui evidentemente aumentano i costi che saranno sostenuti dall'apparato giudiziario in funzione di questa innovazione; presenta quindi un problema di compatibilità tra la vecchia copertura ed una nuova ipotetica copertura in relazione all'ampliamento della platea. È un'obiezione estremamente strategica e fondata. Invito pertanto la Commissione

L'amministrazione penitenziaria deve organizzare corsi di preparazione al rilascio per i condannati che devono scontare meno di sei mesi di pena residua. Essi vanno organizzati in concorso con gli enti locali e con le organizzazioni private. A tal fine deve favorire la presenza di questi detenuti in appositi istituti omogenei"».

luogo in cui nascondere tutto ciò che non va bene, una sorta di pattumiera della società, ebbene bisogna immaginare anche il reinserimento dei detenuti. Sappiamo quanto nelle carceri italiane manchi tutto quello che dovrebbe portare alla pena come rieducazione e riabilitazione: mancano gli assistenti sociali, il

che comportava effettivamente una svolta epocale nella lotta alla criminalità organizzata. Sappiamo che è sempre più difficile difficile combattere la criminalità organizzata perché c'è una rincorsa tra i mezzi di investigazione e le cautele prese dalla criminalità organizzata per evitare che si possano trovare prove a suo carico.

31 maggio 1965, n. 575, il primo periodo con il seguente: «Con l'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica».

la criminalità organizzata non fa più di una telefonata dallo stesso cellulare e poi lo butta via, gettando non solo la scheda, come faceva una volta, ma l'intero telefono perché ha saputo, attraverso il deposito degli atti, che la Polizia riusciva a risalire

strumento veramente efficace nei confronti della criminalità organizzata fosse invertire l'onere della prova sulle ricchezze improvvise.

Questa è la domanda che angosciosamente mi pongo, posto che tutti quanti noi sappiamo che una delle cose che sta affliggendo l'Italia è l'enorme evasione fiscale che non permette, anche in questo momento

cioè la risistemazione dei poteri di iniziativa e di seguito nel procedimento di prevenzione del procuratore della Repubblica ordinario e del procuratore distrettuale antimafia. L'articolo 11 è già stato soppresso in Commissione perché le disposizioni in esso contenute si trovano in altre norme del sistema della prevenzione. dal senatore D'Ambrosio trovano risposta nel complesso delle altre disposizioni, mentre quelle relative all'articolo 25 riguardano tutt'altra cosa, cioè la ridefinizione dei poteri di iniziativa della magistratura inquirente in materia di prevenzione.

l'articolo 29 che individua i beni sequestrabili collegati ad una persona imputata di un reato, cioè il sequestro preventivo relativo ai reati. Vengono inseriti, nel caso dell'articolo 29, cioè del sequestro preventivo, le azioni, le quote sociali e i beni finanziari dematerializzati.

deve essere il medesimo anche su azioni, quote sociali e strumenti finanziari dematerializzati. Non capisco perché nei procedimenti di prevenzione antimafia si possano sequestrare certi certi beni e non altri mentre nei processi normali si possono sequestrare preventivamente anche le azioni, le quote sociali e i beni finanziari dematerializzati. È un problema di simmetria

Ecco perché insisto in un voto favorevole di questo emendamento.

che si pone è come far funzionare un'impresa dove lavorano tanti soggetti dimostrando che lo Stato, quando sequestra un'impresa alla mafia, non la fa fallire e non fa perdere occupazione, i lavoratori di tali aziende non hanno nessuna responsabilità del fatto che il loro titolare si sia macchiato di reati. Per questi motivi abbiamo presentato l'emendamento, che prevede la sospensione delle procedure esecutive degli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in in corso da parte di Equitalia, per non aggravare la situazione di queste aziende; contemporaneamente, abbiamo previsto la sospensione dei termini di prescrizione, in modo tale da non pregiudicare gli interessi dello Stato e i crediti erariali che esso può vantare nei confronti di tali aziende.

e cioè quando questi beni diventano dello Stato, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile, poiché lo Stato acquisisce un patrimonio e diventa creditore di se stesso.

Posso ipotizzare che ci sia un motivo di natura contabile, perché lo Stato acquisisce un patrimonio ma perde un credito, ma francamente l'idea che lo Stato diventi creditore di se stesso e che debba continuare ad iscriversi un debito-credito

La Presidenza è orientata ad accettare eventuali proposte di accantonamento su questo ultimo comma. In effetti, preferirei un approfondimento in Commissione bilancio, anche se non mi permetto di entrare nel merito.

è stata già spiegata con estrema chiarezza: in fase di sequestro è irrazionale che un credito erariale possa essere portato a compimento, dal momento che l'azienda - qui stiamo parlando soprattutto di aziende che viene sottratta alla disponibilità dell'associazione mafiosa evidentemente risente di alcuni contraccolpi; per esempio, non può fruire *cash* di flussi finanziari assolutamente leciti. Se a ciò si aggiungesse anche la necessità di pagare immediatamente le tasse si avrebbe la certa decozione dell'impresa stessa. stessa. La prima parte di questa disposizione prevede la sospensione dei crediti erariali, che non pregiudica in alcun modo le entrate dello Stato, perché se l'azienda dovesse essere restituita,

nella fase conclusiva del procedimento di prevenzione patrimoniale, l'azienda è confiscata e a questo punto è irrazionale che lo Stato incameri un bene gravato di imposte che provengono dallo Stato stesso. A conferma di tutto questo, se mi è permesso, vorrei citare alcuni dati che provengono dall'ufficio del commissario straordinario per la gestione dei beni confiscati, aggiornati al 30 novembre 2008. A questa data, risultavano censite, come esito di confisca, 1.130 aziende sottratte alla criminalità mafiosa. Di queste, 315 sono state liquidate;

È un bilancio terrificante, che rischia di far dire ai dipendenti di queste aziende: «stavamo meglio quando stavamo peggio». Ovviamente, non è che il credito erariale è l'unica causa del fallimento della liquidazione, ma almeno

Si tratta cioè di modulazioni della gestione dei beni e di una serie di altre questioni. Mi permetto quindi di sottolineare l'origine documentale dei testi degli emendamenti da noi proposti, nel senso che sono a nostra firma, ma sono

Sì, Presidente.

iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria

anche per le esigenze di polizia giudiziaria e che le finalità possono essere anche di giustizia, di protezione civile e di tutela ambientale. ricompresa nella possibilità di utilizzazione di questi beni tutta quella gamma di ipotesi contenute - in modo certamente più diffuso, ma qui

la norma che ci viene proposta dal Governo presenta sicuramente degli aspetti positivi, ma riteniamo di dover votare a favore dell'emendamento

In particolare, rappresento come si faccia riferimento innanzitutto alle somme di denaro confiscate ed alla loro destinazione e poi alla gestione ed alla destinazione dei beni immobili che devono essere mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile, o che devono essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali al patrimonio, in particolare - lo sottolineo - del comune ove l'immobile è situato, o al patrimonio della Provincia o della Regione. Questo è un aspetto particolarmente importante anche nell'ottica complessiva - mi limito ad accennarlo dell'impostazione federalista, materia che stiamo affrontando in questo momento in altra sede. Inoltre, per quanto riguarda i beni aziendali, in particolare si prevedono una Non viene assolutamente eliminata l'impostazione del Governo, perché la parte finale dell'emendamento riproduce sostanzialmente, anzi quasi alla lettera, la norma proposta dal Governo e dalla maggioranza; quindi,

sottratti alla criminalità,

di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Riguarda, in particolare, la materia della prevenzione di infiltrazioni mafiose in appalti pubblici, tali da introdurre l'obbligo di denuncia di tentativi di estorsione o condizionamento fra i requisiti di ordine generale. Ne consegue il correlativo adeguamento del regolamento e dei capitolati di lavori pubblici, servizi e forniture. Con l'emendamento 32.100 si introducono altresì misure tese a garantire che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e subaffidamenti siano effettuati tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione, con esclusione di cessioni del credito o del debito a terzi sotto qualsiasi forma e di pagamenti con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori ad euro 2.000, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, si dispone l'esclusione dell'aggiudicatario dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante, potendosi anche richiedere, quale sanzione di natura civilistica, la risoluzione dei contratti di affidamento e di subaffidamento. È del tutto evidente che l'approvazione di una norma di questo genere

gli emendamenti da noi presentati sono finalizzati a rafforzare la tutela degli appalti dalle infiltrazioni mafiose.

Quindi devo solo fare affidamento sul prosieguo dei lavori che riguardano il testo unico delle misure di prevenzione antimafia, ossia sul nostro disegno di legge che già pende in Commissione giustizia. sperando di ottenere ascolto anche dalla maggioranza, dei temi estremamente caldi, che riguardano l'infiltrazione mafiosa nel sistema degli appalti. Comunque, insisto per l'accoglimento degli emendamenti.

perché ad avviso del Governo prevede una norma che segna una svolta non soltanto dal punto di vista giuridico, ma anche, se mi è permesso, politico e culturale nel modo di affrontare un tema che è stato sollevato negli ultimi mesi da svariati addetti ai lavori. Penso, per esempio, alle prese di posizione di Confindustria siciliana. Il tema è quello della sanzionabilità

il problema di come dare seguito alle preoccupazioni sollevate, non soltanto da queste fasce coraggiose di industriali presenti in zone a rischio, ma anche dall'associazionismo antiracket e dall'autorità giudiziaria maggiormente impegnata su questo fronte. Abbiamo cercato di evitare una norma che fosse soltanto velleitaria e quindi colpisse in modo indiscriminato tutti gli operatori economici, rappresentando in questo modo una bandierina senza esiti concreti apprezzabili. Abbiamo altresì cercato di evitare l'inserimento di un'ulteriore norma penale, che sarebbe andata incontro alle difficoltà dei vari gradi di giudizio e quindi avrebbe avuto un esito a distanza di molti anni rispetto all'accadimento. Per questo si è immaginato di circoscrivere l'area di interesse quella degli imprenditori che vincono una gara di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici. Costoro hanno un obbligo in più, a nostro avviso, di lealtà nei confronti dello Stato e delle istituzioni. Per questo viene richiesto loro, non un atto di eroismo ma un seguito concreto di questa lealtà, posto che non denunciare richieste estorsive che si inseriscono in un contesto mafioso

alla conclusione di indagini, il pubblico ministero contesti, nei confronti di altri evidentemente, un reato di estorsione o di concussione con l'aggravante mafiosa (articolo 7 del

che questa richiesta di estorsione non è stata denunciata dall'aggiudicatario di un appalto pubblico, parte una segnalazione all'autorità degli appalti, la quale la pubblica sul sito del proprio osservatorio. Dalla pubblicazione sul sito deriva come conseguenza l'interdizione fino a tre anni dal conseguire nuovi appalti pubblici; il che significa - lo ripeto - evitare

operativo a quel gesto di coraggio a cui le istituzioni, in questo caso il Parlamento a cui il Governo affida questa norma, non possono certamente fare mancare una risposta altrettanto concreta e operativa. Proprio perché riteniamo che questa disposizione sia tutto sommato un punto di equilibrio rispetto alle esigenze sollevate e alla necessità di non gravare ulteriormente sull'autorità giudiziaria,

ad una svolta nel prendere in esame la storia e i risultati che si sono ottenuti in questi anni sul versante dell'antiracket con il contributo preziosissimo e insostituibile da parte delle associazioni antiracket. Da più parti ci è stata chiesta una svolta; da più parti ci è stato chiesto un gesto finalmente di grande maturità da parte del Parlamento: fare in modo che di fronte alla richiesta estorsiva dell'organizzazione mafiosa non ci sia più la sola volontà soggettiva, discrezionale e per molti versi fragile degli imprenditori nel dire no, ma ci sia un supporto normativo. Il conflitto tra l'imprenditore che non vuole pagare e l'organizzazione mafiosa con tutta la sua forza e con tutta la sua capacità intimidatrice

interessi forti da parte del mondo dell'impresa, che non solo ha una motivazione ideale nella libertà di mercato di non pagare o una motivazione nella propria dignità di imprenditori, ma anche un interesse forte, consistente nel dire no e resistere grazie alle norme adottate nei confronti dell'organizzazione mafiosa. Il Governo ha preso un indirizzo che a nostro avviso sicuramente va nella direzione degli emendamenti che abbiamo proposto, ma nello stesso tempo però non fa il salto di qualità fino in fondo; una sorta di paura. Le proposte che noi avanziamo, Presidente, non sono quelle di dire semplicemente che chi paga il pizzo

chi paga viene penalizzato, chi non paga viene sostenuto. Questa nostra scelta, signor Presidente, aggiunge un ingrediente potentissimo per disarticolare non più semplicemente

resistendo e denunciando, possono ottenere vantaggi. Sul tema dei vantaggi il Governo si è bloccato e questo è un limite.

inseriamo l'obbligo di denuncia per tutti gli operatori economici. Le penalità - sempre di carattere amministrativo - vanno in capo al rapporto che gli operatori economici hanno con l'ente pubblico, sia

Presidente, in ordine a questa vicenda credo che lei sia perfettamente a conoscenza di ciò che è accaduto in questo periodo nella nostra terra. Ci sono stati risultati positivi, nonostante ciò non vi è ancora una presa di coscienza che possa determinare una svolta. Credo, pertanto, che questo provvedimento, come anche questo emendamento, vadano in questa direzione. Le cito un esempio: dopo gli arresti dei grandi boss e le ultime retate,

Ebbene, questo emendamento e questa scelta potrebbero determinare una svolta, che consiste nel fatto che l'imprenditore non deve scegliere la convenienza, ma deve scegliere lo Stato contro la criminalità,

al fine di consentire una fase di risveglio economico che non soggiaccia più ai voleri della criminalità organizzata. Questo è un modo per dare un contributo forte anche dal punto di vista culturale ad una scelta che in questo momento gli imprenditori spesso non fanno perché sono ricattati ed hanno paura. Basta leggere i giornali di oggi per capire che le tariffe sono scontate, ma nonostante tutto ancora sulle estorsioni la cassa della criminalità organizzata, le casse e i conti correnti dei criminali. Ecco perché in questo momento è importante, proprio adesso, dare un segnale unico da questo Parlamento.

continuo ad essere convinto che la soluzione che viene proposta e che già è stata condivisa dalle Commissioni sia quella di maggiore equilibrio. ancora una volta, in particolare, l'emendamento presentato dal senatore Lumia, che reca anche tante altre firme. si fa stato, per procedere poi all'intervento sanzionatorio, su un accertamento giudiziario che abbia un carattere di plausibilità e quindi la conclusione dell'indagine nel momento in cui il pubblico ministero si appresta a chiedere la citazione in giudizio; invece nell'emendamento del senatore Lumia si fa riferimento ad un accertamento del prefetto,

colui che denuncia il *racket* subisce danni anche «semplicemente» da intimidazione ambientale, non ci sentiamo come Governo di condividere una sorta di premio per l'adempimento di un dovere civico che dovrebbe interessare tutti i cittadini, quale l'obbligo di denunciare l'intimidazione di tipo mafioso, anche perché un'ipotesi di questo tipo si presterebbe inevitabilmente ad usi strumentali, come accade già adesso per alcuni istituti di carattere risarcitorio.

Oggi la certificazione antimafia, così come è strutturata, finisce per essere un peso insopportabile per le aziende

Nell'anno passato il FORMEZ ha svolto su questo argomento una ricerca molto seria e approfondita, tra l'altro con il pieno coinvolgimento delle prefetture di Roma, Napoli, Palermo e Catania,

una scuola che evoca il nome di una vittima della mafia, componente della scorta del compianto giudice Borsellino. *(Generali

del provvedimento ed il successivo articolo 34 tratta un argomento estremamente delicato, che è strategico per la lotta alla criminalità organizzata.

tecniche e giuridiche adeguate per gestire non tanto e non solo i beni mobili ed immobili confiscati alla mafia quanto soprattutto i complessi aziendali che hanno bisogno, per definizione e per struttura,

pertanto, con questi emendamenti, un cambio di rotta sostanziale che riguarda la gestione dei beni confiscati ed una disciplina

e sociale. Quando si confisca un'azienda o un'impresa e non si garantisce la continuità manageriale in termini di efficienza di quella stessa impresa ma se ne dichiara il fallimento in via anticipata, creando crisi di livello occupazionale, si inserisce un corto circuito nel rapporto con la società. Infatti, a fronte di un'impresa mafiosa confiscata, i suoi lavoratori, in buona fede,

ciò che cambia è l'ottica con cui si affronta il problema. Il Governo continua a mantenere una funzione centrale all'Agenzia del demanio, mentre noi riteniamo che il problema della gestione

ritiene infatti che la competenza sui beni è del demanio, ma per la destinazione è competente il prefetto: è chiaro che arriveranno a litigare, perché la proposta deve provenire dall'Agenzia del demanio. Riteniamo che i nostri emendamenti portino

come Partito Democratico abbiamo presentato una serie di emendamenti riguardanti: il riordino della disciplina in materia di misure di prevenzione (il 33.101,

Peraltro, di fronte ad una materia così delicata e, soprattutto, tecnicamente complessa ci è stato proposto in data di ieri dal rappresentante del Governo un ordine del giorno, al quale saremmo intenzionati ad aderire, ritirando gli emendamenti, però con l'impegno preciso di tenere conto del lavoro svolto unanimemente dalla Commissione parlamentare antimafia nella precedente legislatura, che mi sembra aver prodotto anche una relazione finale.

di un accoglimento dell'impegno da parte del Governo a promuovere in tempi brevi una disciplina complessiva sul tema dell'assegnazione e della gestione dei beni confiscati. L'emendamento 33.0.101 (testo 2) interviene in particolare sulla fase di gestione disponendo la costituzione di un fondo a supporto delle imprese interessate in qualità di assegnatarie sui beni confiscati. questa mattina più volte richiamate, queste imprese si trovano il più delle volte ad intervenire su beni in grave stato di deterioramento che richiedono ingenti investimenti perché, nelle more dell'assegnazione, queste aziende non sono gestite, di fatto, e quindi il loro e quindi il loro patrimonio si deteriora. I soggetti assegnatari si trovano spesso nella difficoltà di reperire fondi per realizzare gli investimenti necessari a far ripartire la produzione e quindi la costituzione di un fondo a garanzia di questi investimenti, di un fondo a garanzia di questi investimenti, purtroppo spesso necessari in presenza di interventi delittuosi che realizzano danneggiamenti dolosi nei confronti delle produzioni di tali imprese, è misura indispensabile indispensabile per far sì che il recupero all'economia legale di questi territori e di queste attività sia effettivo e non meramente nominale. Per questo l'invito al Governo ad intervenire presto ed efficacemente su questa materia è davvero caloroso.

ci sono diversi organi che se ne stanno occupando da tempo, oltre alla magistratura, ma con risultati spesso scarsi e talvolta inconsistenti. Riteniamo sia giunto il momento di porre chiarezza, dando consistenza all'organizzazione di un patrimonio che sta diventando sempre più vasto e quindi particolarmente interessante ed utile per il contrasto al crimine organizzato. vada data vita ad un organismo di vertice, sotto il controllo politico della Presidenza del Consiglio dei ministri, che dovrà provvedere, entro novanta giorni, con decreto.

a quello attuale (anche se ancora, da parte della maggioranza, a mio giudizio, non c'è quell'attenzione che meriterebbe una riforma di tal genere nel settore giudiziario). Questa banca dati, Questa banca dati, che, ripeto, è una risorsa esistente e funzionante, dovrà essere posta anche a disposizione di tale organismo e, attraverso una cognizione sistematica, si potranno evitare tutte quelle disfunzioni, quegli errori inutili e dannosi che riguardano il settore del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata. Quindi, in sintesi, un organismo centrale sotto la responsabilità politica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvarrà sul territorio delle risorse che fanno capo alle prefetture, con l'utilizzo importante della base informatica che già esiste e che va posta al servizio di tale organismo.

il parere contrario

del senatore Saltamartini e 33.106, di cui sono primo firmatario, ma che è stato illustrato dal senatore Maritati,

33.101 (testo 2) è stato trasformato in ordine del giorno già accolto dal Governo.

di ciascuno dei suddetti emendamenti. Perciò, se ci sono altre motivazioni sarebbe interessante conoscerle, ma sulla base del tenore letterale di queste disposizioni risulta difficile capire perché vi sia il parere contrario

Grazie

alla compressione di un diritto costituzionalmente garantito quale quello della libertà di riunione. Mi domando pertanto se si tratta di una norma funzionale ad un obiettivo specifico, quale può essere il contrasto al terrorismo, nel qual caso, così come è avvenuto con altre norme che sono state introdotte nell'ordinamento, verosimilmente dovrebbe avere una sua dimensione eccezionale e temporanea. Vorrei capire dal sottosegretario Mantovano qual è la finalità concreta quanto la discrezionalità in capo al Ministro dell'interno nell'attività di scioglimento di associazioni è abbastanza ampia. Credo

Signor Presidente, ringrazio il senatore D'Alia per aver fornito questa occasione di chiarimento. La norma che si intende introdurre su iniziativa del Governo parte da una situazione di fatto

si occultano all'ombra di ONG o, comunque, di sigle associative apparentemente neutre.

salvo poi, all'esito di un giudizio in cui ciò risulti dimostrato, arrivare, se ne sussistono i requisiti, allo scioglimento della medesima associazione. è sufficiente che vi sia un procedimento penale in corso. Ovviamente al Ministro dell'interno, che è autorità nazionale di sicurezza, questo procedimento deve essere comunicato: da ciò la previsione di una comunicazione da L'unico elemento procedurale differente rispetto alla legge Mancino è che il potere di sospensione viene individuato nella titolarità del Ministro dell'interno

che può permettere di evitare il pregiudizio di altre indagini o di altra attività di prevenzione in corso. Quindi, l'obiettivo di questa norma è quello di potenziare lo sforzo di prevenzione da parte delle autorità di sicurezza utilizzando una struttura che è già patrimonio del nostro ordinamento da oltre quindici

L'articolo 33 del disegno di legge riguarda la lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Ora viene introdotto questo articolo aggiuntivo che fa riferimento a tutt'altra fattispecie,

politico-sociale. Il rappresentante del Governo ha detto poco fa che è stata adottata la struttura della legge Mancino.

debba essere adottata integralmente, perché si toccano diritti fondamentali che riguardano la libertà della persona, la libertà di riunione, i diritti di difesa. Quindi, va benissimo che ci sia un'attività Grazie dice che dopo deve intervenire, a seguito di richiesta del procuratore, il tribunale, anche in sede cautelare, in tempi molto rapidi per disporre la sospensione.

espressa dal Governo siamo d'accordo. Non siamo d'accordo sui mezzi che vengono indicati. Per questo abbiamo proposto una serie di emendamenti. Alcuni hanno ricevuto un parere favorevole. però, non a caso quelli fondamentali, cioè quelli che tendono a portare il controllo e far disporre la sospensione di queste attività in capo all'autorità giudiziaria, del tribunale, hanno ricevuto un parere negativo. Così come sugli elementi che devono essere utilizzati per arrivare a questa decisione. Chiediamo di pensarci e di adottare integralmente la struttura della legge Mancino.

il parere favorevole all'introduzione di questa struttura.

d'altra parte si vede nettamente che ci sono nuovi oneri di funzionamento della struttura. È difficile che nuovi oneri di funzionamento non comportino

il presidente Azzollini era fuori dall'Aula quando abbiamo iniziato la discussione su questa vicenda. Parliamo di una struttura che già esiste nell'ambito della Presidenza del Consiglio e che viene finanziata con le dotazioni ordinarie della stessa Presidenza, sia pure come figura di commissario straordinario. Siamo già al primo rinnovo; quindi si tratta di rendere ordinario ciò che è straordinario finora, ma con le medesime dotazioni.

è stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri». In sostanza, l'emendamento parla di una nuova struttura e difficilmente le nuove strutture non costano. Mi pare molto difficile.

Soltanto una relazione tecnica predisposta adeguatamente, che mostrasse che la vecchia struttura si trasforma (probabilmente modificandone la base legislativa o almeno regolamentare) in funzione del conferimento delle risorse che oggi finanziano la vecchia per finanziare la nuova avrebbe indotto un altro argomento. Ma così stando l'emendamento, sulla base del parere del Ministero dell'economia non vedo come potessimo dare un parere diverso da quello che abbiamo

vedo consumarsi un confronto estremamente interessante e costruttivo tra maggioranza e opposizione. Vi sono delle idee diverse, ma sostanzialmente si condivide con grande senso di responsabilità l'esigenza di occuparsi di questo tema anche con la dovuta speditezza. Il timore della Il timore della Presidenza è che approvare un emendamento con il parere contrario *ex* articolo 81 possa non soltanto determinare modifiche da parte della Camera, che avrà il sacrosanto diritto di intervenire nel merito, ma

vorrei proprio sin da ora evitare che nel testo trasmesso al secondo ramo del Parlamento possano esserci norme che, sì, potrebbero essere soppresse dalla Camera ma, ove mantenute, potrebbero costituire

Questa è la riflessione che la Presidenza affida all'Aula e che riguarda l'opportunità o meno di approvare un emendamento che, seppur condiviso nel merito, ha

Colleghi, i testimoni di giustizia sono cittadini onesti, lontani dall'organizzazione mafiosa, che rifiutano la cultura dell'omertà, denunciano, vanno nelle aule dei tribunali a compiere il loro dovere di cittadini e da quel giorno, ahimè, per molti di loro inizia una vita a dir poco infernale. quindi ci fosse la massima attenzione su questo tema dei testimoni di giustizia. Presidente, lei sa che molti di loro le hanno scritto: vi sono stati diversi appelli di tanti testimoni di giustizia. A dire il vero, non sono molti, non è una platea ampia: sono circa una settantina. Alcuni di questi testimoni di giustizia oggi vivono in condizioni disperate. Infatti, una volta che per loro finisce il programma a carico dello Stato, che li protegge e mantiene, dopo aver passato mesi ed anni ed anni in un rapporto assistenziale con lo Stato non sono in grado di reinserirsi nella società e nel mercato del lavoro attraverso una attività autonoma, anche perché molti di questi non sono imprenditori.

che sono chiusi nei loro appartamenti in condizioni difficilissime (devono cambiare generalità e vivono con il terrore), senza essere stati nel frattempo inseriti nel mercato del lavoro,

integrare la normativa sui testimoni di giustizia dando la possibilità allo Stato di avere un'arma in più, non obbligatoria

abbiamo nel trattare e nel reinserire i testimoni di giustizia. Possiamo farlo: è una norma che abbiamo già cambiato, perché l'abbiamo già discussa in altri momenti qui in Aula

giustizia ma di persone incensurate, perbene, comuni cittadini che si trovano coinvolti come soggetti che possono dare un contributo positivo ad un'indagine antimafia e di fronte alla scelta di collaborare con lo Stato,

Non stiamo parlando di atteggiamenti premiali da parte dello Stato (che riguardano la collaborazione degli ex appartenenti alle organizzazioni criminali); stiamo facendo riferimento a persone che non devono essere premiate dallo Stato,

di giustizia, quasi fosse uno *status*. Dietro quella parola vi è una valutazione giuridica: dal provvedimento del 2001 soltanto qualora vi sia un comportamento rilevante in ordine alle conoscenze che si hanno,

Signor Presidente, pregherei il Governo di considerare con la massima attenzione l'emendamento 33.0.102 (testo del fatto che nella discussione generale appena conclusasi presso la Commissione parlamentare antimafia il tema della tutela dei testimoni di giustizia ha trovato unanime convergenza sulla necessità di accordare maggiori tutele a persone che, per rendere un servizio alla giustizia, hanno già accettato lo sconvolgimento della loro vita personale e familiare e restano esposti al pericolo di vita. Intuisco che vi sono problemi, che peraltro non mi sembrano insuperabili, di copertura finanziaria; tuttavia credo che, l'estrema delicatezza del tema e per il valore emblematico che avrebbe una decisione unanime del Parlamento in questa materia, tratterebbe di un contributo morale importante nella lotta - ancora aspra e difficile - ai fenomeni mafiosi che tormentano l'intero Paese e condizionano pesantemente lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia.

Abbiamo la grande fortuna di discutere di questo argomento davanti al sottosegretario Mantovano, che della materia si occupa molto bene da anni (sono almeno tre o quattro legislature che il sottosegretario Mantovano se ne occupa anche da deputato).

in una situazione non solo di straordinaria difficoltà ma anche di incredibile precarietà circa il futuro - possibilità di mantenere la propria famiglia, nonché un ruolo e una dignità legate al fatto di esercitare una professione o svolgere un lavoro

sulla vita delle persone stesse, ma anche sulle relazioni che intrattengono con le istituzioni che le seguono. Credo sia davvero opportuna una soluzione di questo genere, che assicura la dignità di un lavoro, una certezza rispetto alle prospettive e che celebra e premia:

nelle quali ci si muove. È una soluzione dignitosa, da Paese moderno, che spazza via non soltanto le preoccupazioni

Su questo, prima di dedicare un cenno all'esame dell'emendamento, vorrei fare una premessa doverosa. Trovo singolare che a scadenze ricorrenti si parli della gestione dei testimoni di giustizia, che certamente ha mille limiti, senza sentire mai il dovere di ascoltare chi questa gestione esercita. valutazioni fornite a tutti i livelli, anche mediatici, sono fatte sulla base di denunce di persone che magari non sono mai entrate nel programma di protezione o che ne sono state estromesse sulla base di

con le dovute garanzie di riservatezza che la Commissione parlamentare antimafia, oggi presieduta dal senatore Pisanu, è senz'altro in grado di dare, a rendere conto della gestione dei testimoni di giustizia con documenti ed atti, anche relativamente a singole posizioni.

la disciplina è cambiata totalmente ed è stato introdotto un vero e proprio statuto dei testimoni di giustizia che rende la posizione di costoro assolutamente diversa, com'è giusto che sia, rispetto a quella dei collaboratori. Questo ha Questo ha comportato che la gran parte dei problemi incontrati si riferissero alla fase antecedente, non tanto per per anomalie strutturali nella gestione, ma nella configurazione giuridica che non tratteggiava questa linea di confine, sicché si scambiava una persona onesta per un delinquente pluriomicida che, in una logica premiale, aveva scelto di collaborare con lo Stato. Ma dal 2001, anche per coloro che sono entrati prima, vi è una totale diversità quanto ad assegno di mantenimento, alloggio e prospettive di reinserimento, quanto alla possibilità - che non hanno i collaboratori ma i testimoni di giustizia - di chiedere l'acquisto da parte dello Stato a prezzo di mercato

di residenza, proprio perché non è giusto sradicarlo. È giusto che lo Stato si impegni nella sua tutela *in loco* anche perché questo, al di là delle scelte dell'interessato, rappresenta una vittoria per lo Stato, che non costringe le persone oneste a trasferirsi. Sono disponibile in qualsiasi momento a rendere conto dettagliato e nominativo di questa situazione con tutte le garanzie di riservatezza, avendo presieduto la Commissione sui programmi di protezione dal 2001 al 2006 e presiedendola di nuovo Grazie in larga parte dei casi giunto a compimento, di reinserimento lavorativo di tanti testimoni di giustizia ma anche, in certi casi, quanto è stato richiesto e quando praticabile, dello sforzo di permettere ad alcuni testimoni di giustizia, che non fossero operatori economici, economici, la cui attività quindi non fosse ricostruibile in altra sede o non fosse tutelabile nel luogo d'origine, per inserire testimoni di giustizia, per esempio, in aziende che lavorano a stretto contatto con la pubblica prestazione. Naturalmente non dirò neanche sotto tortura i nomi di costoro, perché l'esigenza fondamentale, nel momento in cui il programma va a compimento, è che quella persona non sia riconoscibile.

una sorta di canale privilegiato, di corsia preferenziale per entrare nella pubblica amministrazione: questo significa concretamente individuare, sia pure per pochi numeri, una categoria a sé di ingresso alla pubblica amministrazione in deroga al concorso. Questa categoria a sé avrebbe come effetto immediato l'individuazione dei soggetti. Voglio capire come si spiega l'accesso in un ufficio pubblico, non in una azienda, dove si può dire dire ad una sola persona con mille cautele, ma in un ufficio pubblico: come si fa a garantire un accesso che non sia svelabile perlomeno nei termini generali. l'arma in più in questo caso - non è un argomento polemico ma per esprimere nel modo più chiaro - la si dà alla criminalità mafiosa che quel testimone ha contribuito a disarticolare, nel momento in cui lo si indica come colui che lavora in posto. Proprio perché l'argomento è delicato ogni automatismo è deleterio. Il Governo ribadisce in questa sede il proprio impegno massimo alla ripresa di un'attività lavorativa da parte di ogni testimone di giustizia, anche in continuità con quanto fatto finora, quando non vi è un'attività economica a monte che possa essere ripresa come è accaduto, in aziende che hanno a che fare con la pubblica amministrazione) ed è disponibile ad accogliere un ordine del giorno che, riformulando e riprendendo i temi alla base di questo emendamento, imponga al Governo, con periodicità che stabilirete, di rendere conto dell'attuazione di tale impegno nelle sedi più opportune, a cominciare dalla Commissione parlamentare antimafia. Credo che, per onestà, si debba dire con estrema chiarezza che il rimedio proposto, che ha intenzioni lodevolissime, ad avviso del Governo (per carità, discutibilissimo e contrastabilissimo) appare peggiore del male. Per tale ragione confermo la disponibilità nei termini prima enunciati. il tema è estremamente delicato.

confluiscono sull'esigenza di una tutela, laddove il testimone di giustizia dovesse essere assunto in maniera diretta, seppur riservata, nell'ambito della pubblica amministrazione.

Presidente, mi rendo conto della situazione, ma il tema che volevo porre all'Assemblea è di grandissima importanza e di grande urgenza,

senatore Gasparri è sbagliata dall'inizio alla fine, in quanto il Ministro della giustizia ha preso la decisione e la Corte suprema deve ancora pronunciarsi. I tempi saranno lunghi, purtroppo.

Speriamo di approfondirla e di discuterla la prossima settimana. È un tema che ci riguarda come Paese, signor Presidente. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire perché, nel momento che stiamo vivendo, la legge che abbiamo discusso fino a pochi momenti fa, così come opportunamente introduce una serie di reati e comunque modifica l'attuale sistema delle pene, non può non tener conto - e il tema è stato più volte affrontato dai colleghi

avvio di un percorso di rieducazione che deve riguardare i detenuti, se non vogliamo che gli stessi rimangano tali per tutta la vita, nel senso che non viene proposta loro una soluzione alternativa a quella del crimine. Il mio intervento non vuole assolutamente appesantire il già articolato dibattito della seduta di oggi, ma soltanto porre all'attenzione del Senato l'opportunità vorrei dire l'esigenza - che si porti rapidamente in Aula uno strumento che consenta all'Assemblea di effettuare una riflessione sul sistema penitenziario italiano

dei contenuti dell'articolo 27 della Costituzione (in materia di pena non afflittiva, ma rieducativa), sulle condizioni interne alle carceri, nonché sulle motivazioni che hanno indotto il sottoscritto, sin dal

un reato - per il quale il nostro Paese si è impegnato e ha sottoscritto accordi internazionali - che non è presente nel codice penale italiano e che certamente ha bisogno di essere ben perimetrato e individuato per

con la toga, in altri ancora da uomini con il camice bianco; non c'è dubbio che in questo Paese le divise, le toghe e i camici bianchi non siano di per sé garanzia di corretta momento che i delinquenti possono essere in doppiopetto, con il colletto bianco, con la toga, con la divisa oppure con la coppola (perché tali sono se sono delinquenti

la condizione penitenziaria, l'applicazione dell'articolo 27 della Costituzione e il rispetto degli accordi internazionali in materia di introduzione del reato di tortura non possano che essere affrontati insieme per realizzare un unico

e non possiamo ammettere che Battisti possa essere considerato un rifugiato politico. È solo un assassino.

In quegli anni l'attenzione della politica e dei politici italiani, ahimè di tutti gli schieramenti, salvo quello dei radicali, era molto più dedicata alle iniziative, che alcuni definivano e continuano a definire diplomatiche, di Yasser Arafat piuttosto che alla ricerca di una possibilità della pratica di un sionismo non violento che oggi potrebbe quasi sembrare sembrare una sorta di contraddizione in termini ma che invece si può manifestare con la promozione della legalità, della democrazia e dello Stato di diritto, tanto per gli israeliani quanto per i palestinesi; palestinesi che oggi in Israele godono di diritti civili e politici (con tutte le limitazioni che anche Israele, in quanto democrazia, inizia a porre relativamente al loro godimento), mentre invece dubito che possano continuare a godere di quel minimo di finestra di pratica di politica militante non violenta, che è stata concessa loro ad un certo punto negli anni '90, che li ha portati finalmente ad eleggere alcune delle loro cariche, dal punto di vista parlamentare e dal punto di vista esecutivo. se posso emendare l'appello al cessate il fuoco, direi che non soltanto lo lanciamo tutti insieme, come organi dello Stato, ma che ci rivolgiamo alle due parti in guerra, ritenendo ritenendo che quello sia il primo passo per la ricerca di una soluzione e non l'unico obiettivo politico che la Comunità internazionale in queste ore si propone relativamente ad Israele.

vedo, e al senatore Perduca, che hanno richiamato nel dettaglio il fatto che in Aula si fosse in pochi, che in questo caso si tratta di sollecitare l'intervento dell'Aula e del Governo.

rendersi conto di quello che è stato fatto, o attraverso i Resoconti o con Radio radicale o con altri strumenti informatici che sono disposizione di tutti. Il fatto che non ci sia nessuno significa che chiunque è presente in questo momento in quest'Aula. **Mozioni e interrogazioni,